un testo che è stato presentato dal Governo che peraltro è attualmente in vigore e che poi è stato corretto con alcuni emendamenti della Commissione sui quali

si tratta di una materia sulla quale c'è stata un'ampia convergenza in merito a quello che deve essere il regime che regola i servizi pubblici locali

senatrice Donaggio e del senatore Marco Filippi, hanno ricevuto un parere contrario semplice della Commissione bilancio, ma suscitano un problema sul quale so che c'è una disponibilità del Governo, Grazie,

nel dispositivo siano aggiunte le parole «nel rispetto del diritto comunitario», così che si legga: «l'ente affidante può, nel rispetto del diritto comunitario, indicare tra gli oneri da porre a carico del nuovo affidatario il subentro nei rapporti di lavoro in corso».

che, come abbiamo detto, in maniera del tutto impropria è una vera e propria riforma del comparto

non accoglie nessuno degli emendamenti che cercano di inserire il sistema idrico tra le materie escluse dall'applicazione. Se non è questa la volontà, allora si sopprima l'articolo e si torni in Commissione per realizzare la riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di cui siamo proponenti insieme ad altri colleghi della maggioranza e su cui siamo pienamente disponibili.

ma che viene travisata per mantenere di fatto, magari al di là delle intenzioni consapevoli, un meccanismo di gestione del servizio idrico affidato a società *in house*, nominate dagli stessi Comuni che dovrebbero essere l'autorità in materia idrica e che invece utilizzano questi mezzi per aumentare i canoni del servizio idrico,

migliore utilizzazione di questa ricchezza fondamentale. Invocare un'Autorità per l'acqua, che potrebbe essere essere un'indicazione del tutto estemporanea, non ha senso in questo settore. L'acqua è pubblica, rimane pubblica. Altro è il gas, che è privato e rimane privato, altra cosa sono i mezzi pubblici e le autolinee che rimangono private. È un contesto assolutamente diverso. assolutamente diverso. Chiederei quindi alla collega Adamo di trovare argomenti più solidi per negare la necessità che in questa materia, ferma restando la proprietà pubblica delle acque e delle reti, la gestione delle reti e l'erogazione del servizio vengano affidate attraverso gare ad evidenza pubblica per un maggior vantaggio degli utenti.

15.31 e 15.501 puntano a garantire il mantenimento della proprietà e della gestione pubblica del servizio idrico.

proprietà pubblica dell'acqua e sua gestione: è una pura finzione. Se la proprietà rimane pubblica ma la gestione è affidata ad enti separati e privati, l'esito l'abbiamo già sotto gli occhi. Ormai c'è una larghissima pubblicistica di esperienze europee che dimostrano come questa separazione, questo affidamento della gestione ad aziende private determini peggioramento del servizio, aumento smisurato dei costi, sostanziale inaffidabilità dell'insieme. Nella Regione Toscana, da cui provengo, il caso di Arezzo meriterebbe di essere approfondito dai colleghi della maggioranza, perché è il caso pioniere: una città che ha voluto praticare questa scelta, e che oggi si trova di fronte alle conseguenze che dicevo prima, e cioè aumento dei costi, peggioramento del servizio, peggioramento dell'acqua stessa. stessa. Nella gestione di un bene comune - del principale dei beni comuni - come l'acqua non ci si può affidare ad una realtà che poi diventa insensibilmente e progressivamente un assembramento

che peraltro esprimo a titolo personale e che non impegna il mio Gruppo, riguarda la scelta di inserire i servizi idrici tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica. Ebbene, io non condivido questa scelta, non perché sia in via teorica contrario alla possibilità di affidare anche a soggetti privati la gestione dei servizi idrici, ma perché credo che nel caso dell'acqua, un bene comune e non privatizzabile sulla base di innumerevoli norme e principi internazionali, il criterio della gestione non debba rispondere preliminarmente a logiche mercantili. L'acqua non è una merce e quindi non può essere comprata e venduta alla stregua di una merce. Nel merito, anche rispondendo alle argomentazioni che svolgeva ieri il collega Saro, osservo che non si capisce per quale motivo sarebbe ideologica la posizione di chi è contrario alla privatizzazione senza se e senza ma, e invece sarebbe pragmatica la posizione di chi è favorevole a tale privatizzazione incondizionata. Aggiungo anche che, come certo molti colleghi sapranno, è tutt'altro che unanime, anche tra i giuristi, l'opinione che dalle direttive europee che si occupano di servizi pubblici (la direttiva 92/50/CEE, la 93/38/CEE e poi la più celebre Bolkestein) derivi automaticamente l'obbligo di privatizzazione La seconda considerazione, in larga parte già illustrata dalla senatrice Adamo rispetto all'emendamento soppressivo dell'articolo, riguarda l'obiettivo di ridurre il danno delle norme che vengono proposte. Non c'è alcuna ragione di ordine comunitario che giustifichi le previsioni dell'articolo 15. Tale articolo mette in discussione buona parte degli affidamenti effettuati negli ultimi dieci anni, specialmente quelli a società interamente pubbliche, pubbliche, cosiddetti *in house.* Tali affidamenti non solo erano conformi alle leggi vigenti all'epoca ma sono stati valutati legittimi dalla Corte di giustizia delle Comunità europee e recentemente, pochi mesi fa, hanno ricevuto l'approvazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che, con deliberazione dell'aprile di quest'anno, ha riconosciuto la conformità di gran parte degli affidamenti *in house* esaminati alle leggi italiane ed europee. europee. L'emendamento in titolo, come altri che ho presentato, punta a ridurre il danno che questa norma è destinata a recare, evitando in particolare la cessazione anticipata anche delle gestioni affidate, conformemente alle norme comunitarie, e prevedendo specifiche tutele

non ci sono obblighi comunitari né sentenze della Commissione che possano imporre alcuna esecuzione. Con questo provvedimento si dispone la definizione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e si escludono settori importanti come il gas, la distribuzione di energia elettrica e il trasporto ferroviario regionale, nel presupposto che tali attività costituiscano una specifica attività che merita una particolare attività normativa. Dal momento che il servizio idrico integrato è già disciplinato dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalla legge n. 36 del 1994, non si capisce perché non debba risultare escluso, esattamente come si propone di fare per il gas, per l'energia elettrica e per il trasporto pubblico locale. Per questo motivo, sosteniamo l'emendamento 15.84 che esclude da questo intervento il servizio idrico integrato.

non vi è alcun dubbio che la gestione delle farmacie comunali rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica. Qualora, quindi, la maggioranza e il Governo li approvassero dimostrerebbero tutta la loro schizofrenia. Un attimo fa è stato respinto il nostro emendamento relativo alla regolazione dei servizi idrici che avrebbe assicurato una liberalizzazione in questo campo, consentendo però di affermare l'interesse pubblico. Se la maggioranza approvasse questi due emendamenti identici escluderebbe dai servizi pubblici a rilevanza economica le farmacie comunali, quando è del tutto evidente che esse hanno invece una rilevanza economica. È chiaro che le farmacie sono anche un servizio di carattere sanitario, ma vi sono norme di settore che rimangono in vigore e che assicurano la continuità di questo carattere delle farmacie comunali. Sottrarle alla liberalizzazione significa farne impropriamente oggetto di un monopolio pubblico quando, invece, vi sono svariate esperienze che dimostrano che attraverso la liberalizzazione si è potuto mantenere questo carattere di servizio pubblico e, nello stesso tempo, consentire ai Comuni di incamerare risorse importanti. Per questo mi appello anche alla maggioranza affinché questa proposta emendativa venga respinta.

l'attenzione che il Governo intende destinare ad un settore dell'assistenza sanitaria così delicato quale è quello garantito dalle farmacie comunali. ciò è tutt'altro che schizofrenico, anzi, è coerente con tutte le disposizioni vigenti, comprese quelle di rango europeo: mi riferisco alla cosiddetta direttiva che ha escluso queste materie dall'ambito dell'applicazione delle norme sulla concorrenza e sul mercato, e alla recente

all'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992. Credo che l'accoglimento da parte del Governo e del relatore di questo emendamento confermi

Presidente, onorevoli colleghi, semplicemente per dichiarare il nostro voto favorevole al nostro emendamento, che tende ad escludere

c'entra? MAZZATORTA *(LNP)*. ...ha venduto le proprie farmacie comunali ad una multinazionale tedesca. E noi oggi siamo costretti, con l'articolo 20, a risolvere il problema creato dal sindaco di Bologna, che oggi si oppone... MAZZATORTA *(LNP)*. Siamo al paradosso. Escludiamo un settore di grande rilevanza sociale dall'applicazione di una disciplina che deve valere per altri servizi

eleva le soglie di esenzione dal parere dell'Autorità garante l'affidamento diretto avrà ancora più spazi. Quindi, vi invito a leggere con attenzione le norme e, soprattutto, gli emendamenti.

Anticipano i soldi allo Stato e garantiscono un servizio pubblico. Le farmacie si sono anteposte a quei vuoti che lo Stato pone in essere creando le condizioni a che i grossi depositi farmaceutici, soprattutto nel Meridione, si appropriassero, con un sistema mafioso, della proprietà delle farmacie, visto che gli altri non pagano, visto che le farmacie si sono indebitate fino al collo. Ecco allora

un nostro assenso. Per questo motivo, sono contro le valutazioni del senatore Vitali.

Come si fa, di fronte all'opinione pubblica, a non escludere l'acqua, bene universale prezioso, e a tutelare le regole, fuori dalle norme europee, per la vendita delle farmacie comunali? stimabilissime *lobby* dei farmacisti sì, i cittadini no. Questo è il messaggio che esce!

Grazie, senatore Cursi.

semplicemente per dire, signor Presidente, che con questo emendamento si conferma tutto ciò che è stato sostenuto dalla maggioranza, e cioè che i servizi pubblici rimangono saldamente nella titolarità e nel governo

noi affermiamo tale principio non solo per i servizi e per le risorse idriche, ma anche per gli altri servizi pubblici locali. Dunque, esso ci sembra perfettamente coerente con le dichiarazioni della maggioranza, se fossero sincere.

Il collega Pastore, replicando alla senatrice Adamo, ha detto che l'acqua è pubblica e rimane pubblica, se ho compreso bene. Dunque, la risorsa idrica è pubblica e le reti rimangono pubbliche. Aggiungo che la Costituzione affida la titolarità della gestione delle risorse idriche alle Regioni. Con questo emendamento noi affermiamo tale principio, quale che sia la forma di gestione che le leggi di settore definiscono. Per questo motivo ci sembrerebbe ovvio che venisse approvato.

senza che nessuno si esprima in modo compiuto e senza che il Governo esprima una posizione chiara. Rispetto all'emendamento 15.504 (ed è questa la ragione del mio intervento),

della natura di bene pubblico della risorsa idrica; quindi, si sta ponendo un argine alle operazioni che le istituzioni locali nel caso possono effettuare. Vorrei capire se il Governo

appalti trasparenti e gare aperte a tutti con regole precise, dettagliate e stringenti e dove il titolare del bene, che è un soggetto pubblico, compie il suo dovere di controllore, verificando cioè che il servizio venga svolto secondo i canoni e i criteri fissati nell'atto di assegnazione del servizio

attraverso una società *in house* costituita dagli stessi amministratori del consorzio dei Comuni responsabile del servizio idrico,

necessarie e sottintese, ma molto spesso espresse dal nostro sistema in questa materia ed, in genere, nei servizi pubblici quando vi è un bene che viene

abbiamo riscontrato come tutte le cosche siano interessate al bene dell'acqua. Per decenni o meglio per centinaia di anni i briganti ed i mafiosi hanno utilizzato questo bene per arricchire le proprie casse e per far soccombere i cittadini normali.

che sono un bene essenziale! Vi state macchiando ancora una volta di una scelta errata! Presidente, risparmio osservazioni che hanno già svolto altri colleghi sul fatto che questa materia venga trattata in un decreto-legge, peraltro con una pertinenza rispetto all'oggetto del decreto che è tutta discutibile. Mi rivolgo Mi rivolgo al senatore Pastore innanzitutto, ma anche agli altri colleghi: quella che riguarda la gestione di una risorsa come l'acqua non è una questione

Sembrerà paradossale ai colleghi che vorrebbero procedere con una certa rapidità, ma questa è una questione sulla quale si interroga il mondo, cioè è una delle grandi questioni sulle quali il mondo intero, Governi, associazioni, popoli si interrogano. Non è quindi questione di poco momento, e non possiamo pensare di tirare innanzi come se niente accadesse. Stiamo Stiamo discutendo di una questione essenziale, che è, devo dire, felicemente sintetizzata nell'espressione che hanno adoperato i colleghi, e cioè dell'accesso universale alla risorsa costituita dall'acqua. Ovviamente, ogni qualvolta discutiamo di accesso, discutiamo di una quantità di questioni che erano, nell'emendamento che avete respinto, puntualmente enumerate (e probabilmente alcune ne mancavano); questioni sulle quali, ripeto, le grandi agenzie internazionali si interrogano. Allora, poiché penso ci sia con una consapevolezza diffusa tra i colleghi dell'importanza e della delicatezza della questione, accantoniamo questo emendamento, torniamo a ragionarci, compiamo una verifica puntuale della legislazione, cerchiamo di capire se e come questo emendamento possa completarla o se, come sostiene il senatore Pastore, sia assolutamente inutile e superfluo. Credo che lo dobbiamo alla delicatezza

cattiva, addirittura pessima, e non deve spiegarmi quali sono le esigenze che muovono, nella gestione di alcuni servizi pubblici o anche di beni pubblici, ad aprire ad un mercato trasparente. Ma dobbiamo avere l'attenzione derivante dal fatto che stavolta stiamo parlando dell'acqua, cioè della risorsa in assoluto più preziosa, naturalmente a disposizione dell'umanità.

i servizi pubblici a carattere non commerciale e ad obiettivo sociale non possono essere qualificati e ricompresi tra i servizi di interesse economico e di conseguenza non possono essere soggetti alle regole del mercato interno». posto in votazione perché accolto dal Governo. Il Governo è in contraddizione, avendo presentato l'articolo 15. Presidente, qual è il valore degli ordini del giorno approvati in Aula? Non parteciperò al voto finché ciò non mi sarà spiegato.

il voto in dissenso dal Gruppo, annunciando che non parteciperò alla votazione, come forma di protesta nei confronti di un metodo che viene assunto e che riguarda il fatto che su una riforma di grande rilievo, quale quella dei servizi pubblici locali, ancora una volta si interviene con un decreto

ho ben presente la distinzione esistente tra la proprietà delle fonti idriche e la possibilità di gestire reti che

Neanch'io parteciperò al voto. Chiedo al Governo semplicemente di prendere in considerazione sul serio la richiesta che la presidente Finocchiaro ha avanzato. Di fronte ad un tema così importante, cruciale e delicato, quando tutta l'opposizione vi chiede di accantonare per un approfondimento un emendamento e di tenere aperto uno spazio di dialogo, questa chiusura e questa

ed occorre facilitare l'accesso delle piccole imprese creando nell'ambito della normativa nazionale condizioni di accessibilità migliori per le stesse». In questi due emendamenti si cerca di far sì

Presidente, in questo momento scrivere la norma in un modo ed avere un ordine del giorno che prevede parametri diversi rischierebbe di essere contraddittorio. Bisogna vedere come

auspicata da chi, negli anni scorsi, ha raccolto quasi mezzo milione di firme per evitare che l'acqua venisse privatizzata. Suggerisco al senatore Sangalli, che sta preparando il suo ordine del giorno, che sostengo, di tenere in considerazione - lo stesso invito rivolgo alla maggioranza - il fatto che negli ultimi vent'anni quello dell'acqua è diventato un *business* da 500 miliardi di dollari, che con il passare del tempo è stato attribuito a tre grandi multinazionali. Allora, visto e considerato che avete forzato le procedure ed infilato questa misura all'interno di un'altra che tutto ha a che fare tranne che con i servizi pubblici a livello locale, consideriamo che si può aprire una porta ad una formazione di cartelli transnazionali di megaconglomerati che

sugli specifici settori siano chiamati ad esprimere un parere preventivo sulle deroghe riguardanti gli affidamenti *in house*. Nel caso dell'acqua un organismo di vigilanza già esiste ed è la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche. Non aggiungo ora nulla alle argomentazioni svolte ieri dal senatore Morando sulla necessità di varare una autorità per la regolazione del servizio idrico,

Grazie,

Presidente, il senatore De Sena ha apposto la sua firma agli emendamenti della senatrice Vicari nella formulazione originaria che si riscontra nel fascicolo e solo per questo ha ritirato l'emendamento 15.516. Credo che adesso voglia conoscere la nuova formulazione per poter confermare o no il ritiro dell'emendamento

Prego

che ha bisogno di una adeguata rete di sostegno, in particolare per quanto attiene alle tutele del lavoro. I cambiamenti che si introdurranno produrranno significative ricadute sui lavoratori addetti nei vari settori

sostengano il lavoro. Come in ogni ristrutturazione sono necessari interventi che abbiano anche carattere previdenziale, come pure è opportuno introdurre una parificazione fiscale in materia di IRAP e di deduzioni fiscali e di armonizzazione del costo del lavoro, in maniera particolare per quanto riguarda le aliquote previdenziali. Infine si rende necessario estendere la disciplina della Cassa integrazione guadagni anche in questi settori che ne sono completamente sprovvisti.

Accanto al senatore Comincioli, va bene? Ci sono tanti giornali che capisco siano interessanti, ma coprono una postazione

che è stata inserita finora in tutte le leggi che questo Parlamento ha approvato, che non fa altro che salvaguardare le norme statutarie e degli Statuti di autonomia. È una norma, per la verità, pleonastica, perché comunque le norme statutarie autonomistiche valgono perché sono di rango costituzionale. Ma purtroppo la legislazione italiana ha richiesto, nella sua esecuzione, queste clausole per evitare che le

15.600 è stato ritirato.

modificato nel senso che l'impegno del Governo sia a valutare l'opportunità di autorizzare la detrazione di cui si parla nell'ordine del giorno. Il senatore Mazzatorta fa cenni di assenso,

Vorrei esporre qualche considerazione nel tentativo di farlo recedere da tale invito e, se possibile, di sollecitarlo ad esprimere un parere favorevole, per ragioni molto semplici. L'emendamento da me presentato tende ad imporre l'obbligo dell'indicazione *«made in»*. È vero, me ne rendo conto, che nella relazione al decreto sono state espresse le motivazioni secondo le quali è necessaria, per conformarsi ad alcune pronunce della Corte di giustizia delle comunità europee, la non indicazione «*made in*». Ciò per favorire l'integrazione, ma con una

il prodotto nazionale. Trovo tale motivazione assolutamente incongrua e soprattutto in contrasto con quanto prevedono altri trattati internazionali di pari efficacia rispetto a quello di Roma. Non dimentichiamo che, se dobbiamo fare una gerarchia delle fonti, anche alla luce di quanto dispone

con lo spirito della produzione e soprattutto tenda a recuperare la tradizione e a conservare la fama di

Colleghi, per cortesia.

(in questo momento in una fase di sostanziale blocco a Ginevra, ma che si sono sviluppati prima a Cancùn e poi ad Hong Kong, dove ero presente)

al Governo, ed è stato seguito dai vari Governi che si sono succeduti con la massima decisione. Ricordo in modo particolare l'azione decisissima che fu dispiegata

a tenere un atteggiamento forte, vincente e determinato - naturalmente non solo come Italia, ma nell'ambito di un concerto comunitario - per far sì che il Commissario europeo al commercio possa farsi valere a Ginevra per sostenere questo punto di vista,

Senatore Sangalli,

Per questo motivo, vorrei dirlo chiaramente, sottoscriviamo l'emendamento 16.500. Vorremmo sostenere tale emendamento

però anche dire che le parole, sagge e illuminate, del senatore Scarpa Bonazza Buora mi hanno indotto e mi inducono a riflettere e a fare della prudenza, quella che gli antichi chiamavano *auriga virtutum,* la mia stella polare in questo momento. Vorrei però rivolgere un invito all'Esecutivo. Il Governo sa benissimo che non parliamo più di un mercato europeo, né di una sorta di primazia dell'Europa ci muoviamo e convergiamo in un mercato globale. Il rifarsi ancora a certe pronunce giurisprudenziali che cercano quella integrazione europea, che sicuramente non può essere trovata attraverso questi mezzi ma attraverso mezzi politici, finanziari ed economici, può essere uno strumento forte: ciò deve costituire un impegno da parte del Governo a perseguire tale finalità. È una finalità che per l'Italia è importante e prendo atto con grande piacere che questo sentimento è comune a tutta l'Assemblea.

vorrei sottolineare la valenza dell'articolo 16 che noi approviamo *in toto* e che tende a porre fine a quella che è diventata una moda ed una consuetudine:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 17.0.1/1, 19.0.503, 20.0.505 e 20.0.506, nonché parere di semplice contrarietà sulle proposte 19.0.500 (testo 3)/106 e 17.0.1/2. Esprime poi parere non ostativo sulla proposta 19.0.500 (testo 3) a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che sia soppresso il comma 25. il parere di semplice contrarietà è reso con la segnalazione che l'approvazione di una

"L'assenso del proponente, necessario alle aggiunte di firma di emendamenti, è normalmente presunto, salvo tempestivo, espresso diniego. In caso di ritiro da parte del proponente, gli altri firmatari possono mantenere l'emendamento, in conformità della disposizione di cui all'articolo 102, comma 6, del Regolamento, che consente a tutti i senatori di far propri gli emendamenti ritirati. Conformemente alla prassi, quando il proponente ritira un emendamento per trasformarlo in ordine del giorno ai sensi dell'articolo 95, comma 7, del Regolamento, gli altri firmatari non possono

solo far rilevare che ricordavo bene: nel momento in cui si aggiunge la firma e si fa proprio l'emendamento, esso non è più disponibile solo per il presentatore.

questa mezza misura aggiunta alla decisione cui lei ha fatto riferimento, di cui comunque prendiamo atto, sollecitandone la modificazione per il futuro.

c'è un invito al ritiro

riferisco alle fibre seriche, un'eccellenza per l'Italia. La produzione nazionale di filatura non esiste più già da diversi anni. Questo significa che la produzione tessile, in questo caso quella comasca ma anche nazionale, può essere esclusa dall'attribuzione del «*made in*»*.* Rischiamo di perdere un'eccellenza, sotto questo punto di vista - lo dico anche al relatore Malan - ed è un esito paradossale che francamente facciamo fatica ad accettare: lo accettiamo solo perché sappiamo che il ministro Ronchi è fattivamente impegnato in sede europea su questo argomento. Riteniamo pertanto urgentissimo che il Ministro prosegua la sua attività persuasiva nei confronti dell'Unione europea e che si riprenda con forza questa politica nei confronti di Bruxelles, prendendo slancio dall'attenzione oggi attribuita alla questione del tessile.

il sistema di tracciabilità obbligatorio a livello europeo, al di là delle questioni procedurali che abbiamo sentito poco fa; la riforma delle regole di origine preferenziale; la riforma delle regole di origine semplice. Solo in questo modo daremo un futuro al sistema tessile - e non solo - italiano.

dal senatore Giuliano, diventato ordine del giorno, dimostra che si può essere padroni di un emendamento o di un ordine del giorno ma non della propria politica, perché in quel caso è la propria maggioranza che governa il proprio emendamento o il proprio ordine del giorno.

che ci sono dei dubbi che il censimento dell'agricoltura venga fatto con grande precisione dall'ISTAT. Traduco: sembra che sia un tentativo da parte del Governo in parte di aiutare

nel lavoro e speriamo che poi il Governo abbia il coraggio di essere conseguente alle affermazioni che la maggioranza legittimamente fa e su cui noi concordiamo in Commissione agricoltura.

che consentiranno, se saranno condivise dal Governo e approvate dall'Aula, di superare la convinzione burocratica secondo cui vi sarebbe differenza fra il pescatore professionale - per così dire - tradizionale e il pescatore professionale subacqueo, per cui sono state denegate alcune richieste da parte di questi ultimi tendenti a poter praticare la cosiddetta pesca turismo, cioè la possibilità

si tratta di un settore di economia estremamente limitato, ma non per questo poco significativo in alcune aree del Paese, e mi riferisco, per esempio, alla Sardegna, dove è praticata la pesca del corallo e altro tipo di pesca subacquea. L'università di Cagliari, peraltro, con una proposizione molto meritoria, ha stretto delle alleanze con coloro che praticano la pesca di profondità, in cambio dei reperti che possono essere raccolti intorno ai 130 metri nei 16 minuti in cui dura il periodo di pesca vera e propria, dal momento che le restanti sette ore sono destinate al rientro in superficie. È inutile che spieghi ai colleghi

di un'attività per la quale non è dato alcun contributo, non solo non vi è una maggiore spesa, ma anzi vi è una maggiore attesa di incasso fiscale a fronte di un maggiore reddito da parte degli addetti ai lavori.

il nostro compito sia quello di rafforzare le funzioni dell'ISTAT, a cui sono stati tagliate in modo piuttosto preoccupante le provvidenze e le destinazioni di bilancio. Dunque, solo l'ISTAT deve essere l'autorità statistica di questo Paese.

sostituire un'altra agenzia all'ISTAT nell'organizzazione del censimento generale dell'agricoltura sarebbe un peccato capitale: sarebbe come sostituire la banda d'Affori all'orchestra della Scala.

17.0.1/1. CARUSO *(PdL)*. Allora, non ho interesse e ritiro entrambi gli emendamenti. Non esiste alcuna spesa; la Commissione bilancio versa in evidente errore nel dare questa indicazione.

Ricordo a me stesso e ai colleghi che si sono occupati e si occupano quotidianamente di pesca, per esempio in Commissione agricoltura, che per aggiungere una licenza ad un pescatore che ne abbia già una o due basta un atto amministrativo. Un decreto ministeriale del Ministro o del Sottosegretario delegato, in questo caso,

che intendono accedere alle risorse comunitarie, assume la funzione di una sorta di documento d'identità. C'è poi da dire che l'informatizzazione dei fascicoli può consentire di costruire un sistema informativo ittico nazionale, volto volto alla raccolta e alla condivisione delle informazioni strutturali e durevoli relative a ciascuna azienda operante nel settore della pesca. In conclusione, il fascicolo aziendale è un congegno efficace, a nostro giudizio, dal punto di vista amministrativo per la semplificazione della gestione delle domande di sovvenzione e delle dichiarazioni di produzione dei pescatori e potrebbe anche assicurare il rapido svolgimento dei controlli tecnico-amministrativi, in modo da garantire la conformità del pagamento dei contributi in linea con le norme comunitarie, anche di quelle fissate dagli obblighi comunitari di cui al regolamento 1198 del 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca. A nome dell'intero Gruppo del Partito Democratico esprimo, per questa ragione, voto favorevole.

che desta forte perplessità sia dal punto di vista formale in seguito alla sua difficile applicazione, sia dal punto di vista del merito. Infatti, il presente articolo nasconde, a nostro la solita norma di favore disegnata solo per una categoria di produttori, ovvero i grandi splafonatori, proseguendo così nella logica ormai fatta propria da questo Governo di premiare i disonesti e i furbi a scapito degli allevatori onesti che hanno sempre agito nel rispetto della legalità. Riteniamo, inoltre, che una disposizione come quella recata dall'articolo in oggetto rischierebbe di compromettere fortemente gli equilibri finanziari e di bilancio dell'Agenzia Pertanto, se il Governo avesse voluto adottare una disposizione volta realmente ad agevolare i produttori del settore lattiero-caseario, soprattutto in considerazione del grave momento di crisi che sta attraversando il comparto, avrebbe dovuto provvedere ad adottare un'agevolazione nel versamento del prelievo mensile da parte di tutte le aziende acquirenti di latte e non solo di alcune - individuabili tra i grandi splafonatori provvedendo conseguentemente a coprire il predetto intervento agevolativo con adeguate risorse finanziarie, cosa che non è avvenuta. Poiché la norma in esame ci sembra di tutt'altro tenore ed onestamente non si comprende come possa venire incontro - come sostiene il Governo

affermato il collega Di Nardo, gli emendamenti riguardano l'articolo 18 recante «Disposizioni in materia di prelievo mensile». In sostanza, si tratta delle multe comunitarie che devono pagare gli allevatori di bovini da latte che superano il quantitativo di produzione loro assegnato. Con questo articolo si propone un'agevolazione che ci trova d'accordo nelle sue motivazioni generali, visto il momento drammatico della crisi del settore (in particolare proprio di quello

possono essere utilmente svolti in altra sede per consentire alla collega Pignedoli di terminare il suo intervento. Come dicevo, avendo abolito la legge n. 204, secondo cui chi non versa mensilmente non accede alla compensazione, in questo modo si riammettono anche i grandi splafonatori.

chiede che, se agevolazione vuole essere, venga finalizzata ai produttori in regola, a quelli che accettano di mettersi in regola con gli adempimenti previsti dalle normative, a quelli ubicati nelle zone di montagna

in rapporto alla pericolosità del contenuto dell'articolo 18, in quanto esso mina i princìpi della legge n. 119 del 2003, in particolare quelli del versamento mensile. L'articolo introduce un'agevolazione - il versamento mensile parziale ad esclusivo vantaggio di una categoria di produttori che sono appunto denominati, non a caso, i grandi splafonatori. Non sono prese in considerazione altre categorie, come ad esempio le aziende di montagna e delle zone svantaggiate. Ecco perché, con l'emendamento 18.503 chiediamo che se proprio debba esservi un'agevolazione, magari giustificata dal momento di crisi in cui si trova il settore lattiero caseario in Europa, questa sia rivolta esclusivamente alle categorie di produttori maggiormente esposti alle conseguenze della crisi, ossia quelle aziende che sono ubicate

e voglio ricordare che con la legge n. 33 del 2009 è stato modificato l'articolo 9 della legge n. 119 del 2003 sulla disciplina della restituzione del prelievo versato in eccesso, un articolo che aveva disciplinato la fattispecie con successo e che il Governo e la maggioranza hanno sostituito abbassando dal 20 al 6 per cento la franchigia di splafonamento di chi, essendo in regola con i versamenti delle multe, ha diritto ad eventuali restituzioni di quota che dovessero risultare in eccesso. Parliamo quindi di milioni di euro. Oggi, dopo l'ultimo decreto sulle quote da un lato accade che chi ha rispettato le regole e non ha superato la propria quota ha una tolleranza del solo 6 per cento, e se la supera deve pagare, senza poter accedere alla compensazione nazionale; dall'altro lato, con l'articolo 18

percentuale di splafonamento per accedere alla compensazione. Tale franchigia, che la legge precedente aveva fissato al 20 per cento, è stato abbassato al 6 per cento. Questo limite è assolutamente fisiologico e, come ricordava la senatrice Pignedoli, soprattutto nelle aziende medio-piccole questo 6 per cento equivale ad una produzione lattiera di 15 giorni, facilmente superabile in caso di eventi stagionali appena favorevoli.

debbano essere destinate al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario; un Fondo importantissimo, ma che secondo noi deve essere alimentato con le multe dei grandi splafonatori e non abbassando la soglia di tolleranza al 6 per cento. Sarebbe inoltre assurdo escludere dalla compensazione ed assoggettare alla multa i produttori, in presenza di disponibilità Grazie,

che si riferisce invece unicamente alle società a capitale misto pubblico-privato, anche se con capitale pubblico maggioritario. Si tratta quindi di una precisazione che riteniamo utile per non penalizzare questo profilo di attività. Allo stesso modo, con l'emendamento 19.502 si chiarisce e si cerca di correggere quella che è una pretesa, una imposizione introdotta impropriamente dal Governo e in particolare dal Ministro dell'economia. Ricordo che già due anni fa si erano uniformate le misure e quindi erano partite le azioni di recupero delle somme, come disposto dalla sentenza della Corte, da parte delle aziende che rientravano in quella casistica.

stabilito che le aziende devono pagare interamente tutto il dovuto, anziché consentire una graduazione del recupero e della restituzione delle somme indebitamente riscosse. In questo modo si penalizzano pesantemente i bilanci di quelle imprese. Si crea un danno agli azionisti per le società quotate e soprattutto ai bilanci dei Comuni proprietari di quelle imprese. Aggiungo ‑ non è un elemento di poco conto ‑ che con queste misure si penalizza anche chi è stato più corretto e virtuoso negli ultimi anni, cercando di corrispondere in modo migliore alle indicazioni che la legislazione nazionale chiedeva di seguire per trasformare

In particolare, il terzo comma del nuovo articolo 19-*bis* modifica in un punto essenziale in questa sede abbiamo discusso a lungo e che è stato oggetto di un patto politico tra maggioranza e opposizione, che ha portato tra l'altro anche al nostro voto di astensione.

si cambia quanto previsto nell'attuale legge sul federalismo fiscale, ossia l'obbligo per il Governo di presentare contestualmente al primo decreto legislativo lo schema finanziario relativo agli effetti che la legge ha nei vari territori. Per noi questo è stato sempre un punto fondamentale. Con l'emendamento in esame si sposta il termine al 30 giugno 2010. Si potrebbe ribattere che il 30 giugno 2010 verrà solo dopo qualche mese l'approvazione del primo decreto legislativo, ma da ciò derivano la la nostra preoccupazione e il nostro allarme. In primo luogo, se si cambia già da ora la legge sul federalismo in un punto, la si potrà cambiare anche domani, ed è comunque questa la testimonianza di un atteggiamento elusivo da parte del Governo, e in modo particolare del Ministero dell'economia, già varie volte emerso nel corso della discussione. In secondo luogo, poiché il nostro collega Giulio Andreotti ci invita a pensare male anche se a volte si commette peccato, voglio seguire il suo consiglio. Il nostro Gruppo ha pubblicato i risultati di una simulazione che è stata affidata all'università Bocconi, al centro studi Econpubblica. Risulta che vi sono territori territori che guadagnano e territori che perdono, che non sono però il Nord e il Sud ma territori interni alle grandi aree geografiche del Paese. Allora non vorrei che con questo emendamento la maggioranza volesse evitare di pubblicare tali dati all'approssimarsi delle prossime elezioni regionali, in modo tale da non far capire ai cittadini che non è tutto oro quello che si è promesso, soprattutto in certe zone del Nord. Noi al federalismo fiscale ci teniamo. La maggioranza e il Governo dimostrano di non tenerci quanto noi e per questo sosteniamo il nostro emendamento.

dall'esame del provvedimento in questione. Una Commissione, peraltro, che ha contributo in questi mesi ad orientare non poco l'esito di questo provvedimento. Pur apprezzando, infatti, il concerto intervenuto con le Regioni interessate come il nostro Gruppo chiede da sempre - non possiamo non riscontrare la sistematica procedura elusiva delle prerogative parlamentari delle Commissioni di merito, costrette, anche in questo caso, ad inseguire affannosamente emendamenti presentati all'ultimo momento da parte del Governo, che avrebbero potuto, tra l'altro, ulteriormente giovarsi del contributo delle Commissioni competenti. competenti. Gli emendamenti che abbiamo voluto presentare hanno nella sostanza questa cifra; apportare le correzioni ancora necessarie, che ragionevolmente potevano già essere contenute nel testo e per questo ne chiediamo l'accoglienza al relatore e al Governo. Governo. L'emendamento 19.0.500 (testo 3)/106 interviene sulla proroga dei termini della convenzione vigente, permettendone utilmente la coincidenza con l'anno solare anziché al 30 settembre 2010,

ma la necessità di mantenere delle quote di minoranza societaria; ne individuammo almeno... essere ovviamente anche minore e comunque consentirebbe di monitorare utilmente all'interno il processo di privatizzazione, il cui controllo, purtroppo, per tradizione patria, generalmente cessa con l'affidamento del servizio e l'esperimento della gara. L'emendamento 19.0.500 (testo 3)/110 rafforza il precedente concetto intervenendo, per quanto possibile, sugli assetti societari dei soggetti aggiudicatari del servizio, che noi chiediamo siano tenuti a mantenere inalterati, per almeno cinque anni dalla data di acquisizione, l'assetto organizzativo e l'autonomia finanziaria delle società acquisite, nonché i livelli occupazionali, a prescindere dalla clausola sociale di salvaguardia del personale impiegato che auspichiamo le Regioni inseriscano nel bando di gara. Ricordo che stiamo parlando di marittimi, di lavoratori che non hanno la possibilità di giovarsi dei consueti ammortizzatori sociali.

degli strumenti di cassa integrazione. Nella sostanza, proponiamo il raddoppio dei tempi di estensione da 12 a 24 mesi e, di conseguenza, delle risorse da 15 a 30 milioni di euro.

serve a un'effettiva implementazione delle misure previste dal federalismo fiscale. La Commissione ha iniziato i suoi lavori più

affinché siano contemperati i diritti di difesa dei presunti beneficiari di aiuti illegali o incompatibili con l'obbligo di esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione 19.501, signora Presidente, è volto a garantire il rispetto dei diritti dei contribuenti che potrebbero essere lesi da una previsione che anticipa i termini per il versamento di ingenti somme a titolo di imposte non corrisposte senza collegarvi un'adeguata motivazione. Questa proposta, relatore e rappresentanti del Governo, tende quindi a mitigare l'originaria previsione inserendo due termini per il pagamento, per il capitale oggetto di restituzione da un lato, per gli interessi ad esso afferenti affinché siano contemperati i diritti di difesa dei presunti beneficiari di aiuti illegali o incompatibili con l'obbligo di esecuzione

Grazie,

La Presidenza aveva appena finito di richiamare i colleghi senatori per consentire ai Segretari di Presidenza di svolgere il proprio lavoro.

intervengo per segnalare la resurrezione di una tessera senza la resurrezione del senatore.

Colleghi, per cortesia.

la quale sollecito una risposta. Nel carcere di Brucoli, signora Presidente, c'è un cittadino italiano che da 16 anni circa sconta una pena per un reato... Signora Presidente, poiché la questione che sto affrontando è particolarmente grave, anche se può apparire grottesca, caratterizzata da contenuti estremamente dolorosi, le sarei grato se almeno lei volesse ascoltarmi. dicevo, nel carcere di Brucoli vi è un cittadino italiano che da circa 16 anni sconta una pena per un reato il cui reo confesso è stato già processato, condannato ed ha persino finito di scontare la sua pena.

che, reo confesso, è stato processato e condannato. Il problema è che si è imbattuto in un sistema giudiziario lento, autoreferenziale, poco incline al lavoro, autoprotettivo e costoso, oltre che inefficiente ed ingiusto, che ha provocato questa assurda distorsione. Dunque, c'è un presunto innocente in carcere, mentre il vero colpevole, ripeto reo confesso, condannato per il suo stesso reato, è già libero.

Signora Presidente, oggi abbiamo trovato in casella un *depliant* del Ministero della difesa che ricorda la Festa dell'unità nazionale e giornata delle Forze armate.

www.radioradicale.it, tra gli altri, l'intervento di Marco Diana, maresciallo dell'esercito in congedo, che ha svolto considerazioni sulle affermazioni del Ministero della difesa in risposta all'interrogazione degli onorevoli Villecco Calipari, Schirru e Rugghia sui benefici riconosciuti dall'amministrazione della difesa al maresciallo stesso e ad altri. Ritengo infatti che nel giorno in cui si celebrano le Forze armate si debba tener presente anche

Signora Presidente, la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che condanna l'Italia per l'esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche non si basa di certo su argomentazioni nuove. Nel nostro Paese il crocifisso non è un simbolo esclusivamente religioso, ma culturale e civile. In esso si condensa gran parte della storia italiana e dell'Europa. In esso si riassume una sensibilità diffusa e presente non solo nei credenti, ma anche nei non credenti, in quanto icona dell'amore. Il crocefisso è un simbolo universale, non confessionale. Gli spiriti veramente grandi lo hanno sempre compreso: mi auguro che il Paese Italia rappresentato dal Senato ne abbia un profondo rispetto, come lo ha il popolo padano che mi onoro di rappresentare.

bandito una gara per la raccolta dei rifiuti tossici e particolari. Il dirigente di quell'ufficio è la dottoressa Ferri e la ditta che ha vinto l'appalto è del dottor Ferri. Non so se si

l'uso e l'esibizione di un simbolo della religione cristiana nei luoghi pubblici. Desidero piuttosto intervenire come cristiano o aspirante tale per chiedere che il simbolo principale della religione cui cerco di appartenere non venga usato per fini diversi, che nella teologia cristiana configurano

per il fine di simboleggiare elementi di cultura e di storia di una Nazione equivale a mescolare due piani diversi e a togliere universalità

Grazie,